quarant'anni or sono si compiva con la promulgazione, da parte del Capo dello Stato Giuseppe Saragat, l'*iter* parlamentare della legge n. 300, a tutti nota sotto il nome di «Statuto dei lavoratori». In una difficile stagione politica, segnata da aspri conflitti sociali, dai primi segnali del terrorismo e dal rallentamento della crescita economica, Governo e Parlamento seppero porre mano con decisione all'attuazione di una parte rilevante di quegli ambiziosi obiettivi di tutela del lavoro «in tutte le sue forme e realizzazioni» e di promozione dei diritti sociali e delle libertà sindacali, racchiusi nei Principi fondamentali e nel Titolo III della Parte I della Costituzione. Dal mondo del lavoro e dalle rappresentanze sindacali emergeva con forza l'esigenza di adeguare i rapporti produttivi ai valori costituzionali, considerando il lavoro non alla stregua di una merce da scambiare, ma quale strumento privilegiato per «lo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». La questione di una disciplina legislativa dei rapporti sindacali e dei diritti dei lavoratori all'interno delle aziende, dopo alcuni tentativi falliti nel corso delle precedenti legislature, assunse un ruolo centrale nel programma concordato fra le forze politiche per sostenere la formazione del primo Governo Rumor. Nel chiedere la fiducia al Parlamento, nel dicembre del 1968, il Presidente del Consiglio dichiarò che il Governo considerava prioritario l'impegno di definire, attraverso una legge, una compiuta tutela dei lavoratori all'interno delle aziende, in grado di assicurare «dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro». Alla responsabilità di Ministro del lavoro era stato chiamato l'esponente socialista Giacomo Brodolini, la cui figura si staglia nelle vicende che condussero all'approvazione dello Statuto con i tratti di un vero e proprio eroismo politico e civile. Egli, consapevole di avere la sorte segnata da un gravissimo male, accettò egualmente l'incarico ministeriale in nome di questo obiettivo ambizioso, e dedicò alla sua realizzazione gli ultimi mesi della sua esistenza, consumando in esso ogni residua energia. Gettate le basi della riforma in uno storico discorso tenuto nella città di Avola, Brodolini riuscì, dopo mesi di febbrile attività - della quale anche i suoi più stretti collaboratori ignorarono fino in fondo l'oscura, terribile ragione -, a condurre a termine i lavori di redazione, compiuti da una commissione presieduta da Gino Giugni. Vinte le ultime resistenze di settori delle forze politiche di maggioranza e delle parti sociali, egli portò lo Statuto all'approvazione del Consiglio dei ministri ed alla conseguente presentazione del disegno di legge governativo presso il Senato. Era il 20 giugno 1969. Giacomo Brodolini morirà a Zurigo 20 giorni dopo, senza poter seguire l'*iter* parlamentare del disegno di legge, che sarà condotto all'approvazione delle due Camere dal suo successore Carlo Donat-Cattin. Come affermò Francesco De Martino nel ricordare, venti anni dopo, la figura del suo compagno di partito, l'azione di Giacomo Brodolini e l'approvazione dello Statuto dei lavoratori costituiscono la più chiara dimostrazione che «se c'è una volontà politica, se vi sono degli uomini impegnati» che credono in ciò che vogliono realizzare, non è affatto vero che «il regime parlamentare sia lento ed inefficiente». L'approvazione delle Camere consentì, per la prima volta nel nostro Paese, l'entrata in vigore di un sistema normativo volto a tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e la libertà sindacale nei luoghi di lavoro. Tra le conquiste più significative, la legge ribadisce nel Titolo I, dedicato alla tutela della libertà e della dignità del lavoratore, il riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero anche all'interno dei luoghi di lavoro, introducendo il divieto per il datore di lavoro di indagare sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, in particolare nel momento dell'assunzione, quando è massima la debolezza della parte lavoratrice all'interno del rapporto. I Titoli successivi del disegno di legge, nel disciplinare l'attività dei sindacati all'interno dei luoghi di lavoro, realizzano l'intento di aprire le porte delle aziende alla presenza stabile delle rappresentanze sociali, esercitando (come affermò in seguito Gino Giugni) una vera e propria «azione promozionale» del ruolo del sindacato, per incanalare il conflitto sociale all'interno di forme organizzate in grado di gestire e risolvere le vertenze tra datori e prestatori di lavoro. L'approvazione dello Statuto dei lavoratori e la sua successiva attuazione costituiscono una delle più alte realizzazioni del riformismo politico del secolo scorso. Sulla necessità di conservare e rendere più efficaci le conquiste dello Statuto, di fronte ad un assetto delle relazioni industriali e ad una composizione dello scenario produttivo e del mercato del lavoro in continua evoluzione, si sono misurati, nel corso dei decenni, alcuni fra i più acuti spiriti riformatori del nostro tempo. Essi seppero condurre le forze politiche e le parti sociali lungo un difficile cammino di ponderate e sofferte riforme, che la mano assassina del terrorismo ha voluto, in più di un'occasione, macchiare di sangue, mostrando purtroppo, nel solco doloroso della sua azione delirante, la chiarezza criminale nell'identificare in queste persone e in queste dinamiche politiche e sociali il cuore della modernizzazione del nostro Paese. Penso, in particolare, al grave attentato patito da Gino Giugni, colpevole agli occhi dei terroristi del contributo determinante reso al protocollo d'intesa del 1983 sulla scala mobile, nonché della sua costante opera di riflessione e proposta giuridica in materia di evoluzione del mercato del lavoro e di aggiornamento delle sue tutele. Ma soprattutto penso all'assassinio di Massimo D'Antona, di cui ricorre oggi l'undicesimo anniversario dalla morte, studioso attento dell'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro e pioniere della modernizzazione del pubblico impiego, e di Marco Biagi, portatore del sogno interrotto di una società attiva, nella quale le esigenze produttive potessero finalmente convivere con la qualità della vita personale e familiare del lavoratore e, quindi, con quel pieno sviluppo della persona umana che la Costituzione pone tra gli obiettivi principali dell'azione dei pubblici poteri. Penso a tanti altri sindacalisti, lavoratori, studiosi colpiti da questa violenza criminale, che l'unità delle forze politiche e sociali del Paese ha saputo sconfiggere. Non è questa la sede per interrogarsi sull'attualità delle singole parti di cui si compone lo Statuto dei lavoratori, e sulla sua idoneità a perseguire - nel mondo di oggi - gli alti obiettivi di tutela e di sviluppo umano e sociale che si posero i suoi autori. È certo indispensabile che le forze politiche e sociali si interroghino sui passi necessari per giungere, sulla scorta del pensiero di Marco Biagi, da uno Statuto dei lavoratori ad uno Statuto dei «lavori», al fine di estendere la garanzia a tutte quelle forme di prestazione lavorativa sconosciute al legislatore del 1970, ma divenute ormai preponderanti nell'attuale contesto produttivo, affinché sia assicurata una tutela piena del lavoro «in tutte le sue forme e realizzazioni», come impone la Costituzione. Lo dobbiamo - come sottolinea il costante monito del Capo dello Stato - a tutti quei cittadini in preda alle diverse forme di precarietà del lavoro che, sotto i colpi della crisi economica, troppo spesso vivono in drammatiche precarietà esistenziali. Essi si aspettano dalle istituzioni di una Repubblica fondata sul lavoro una risposta decisa e forte almeno quanto quella data, quarant'anni fa, dai nostri predecessori, il cui ricordo è presente oggi in quest'Aula.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il grande giuslavorista Federico Mancini, in un suo saggio redatto all'indomani dell'approvazione dello Statuto dei lavoratori, scriveva: «Nell'industria italiana, ma soprattutto nei suoi settori più efficienti e tecnologicamente avanzati, gli anni successivi alla svolta del 1948 furono l'epoca della grande controffensiva padronale. Mediante violenze fisiche e morali, controlli, divieti e limitazioni di ogni genere, il movimento operaio fu messo alle corde. La poderosa rete di istituzioni che esso aveva costituito nell'immediato dopoguerra e l'area di potere che si era assicurato nei luoghi di lavoro furono sgretolate e si dissolsero. Le grandi centrali non osarono più proclamare scioperi di portata nazionale, i salari reali persero continuamente terreno. Le ACLI nel 1952, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori del 1959, rivelarono che in migliaia di casi gli attivisti sindacali erano isolati, confinati, licenziati, che i comuni operai e impiegati erano ridotti al silenzio e costretti a subire pratiche umilianti, che le commissioni interne non riuscivano a svolgere i loro pur modestissimi compiti». Scrisse, molto più tardi, Eugenio Scalfari, che in quel decennio regnava incontrastato il «bastone nelle fabbriche». Fu Giuseppe Di Vittorio, al congresso della CGIL tenutosi a Napoli del 1952, a chiedere l'adozione di uno «Statuto dei diritti dei lavoratori». Sosteneva Di Vittorio che non era necessario redigere *ex novo* un catalogo dei diritti fondamentali dei lavoratori; si trattava, invece, di rendere concreto e possibile l'esercizio dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti all'interno delle imprese, individuando le prassi che ostacolavano tale esercizio, reprimendole con un adeguato apparato sanzionatorio. Con felice sintesi si chiedeva di portare la «Costituzione nelle fabbriche». Negli stessi anni Gino Giugni sviluppava, sulla scorta delle sue esperienze di studio negli Stati Uniti, presso l'Università del Wisconsin, un nuovo punto di vista sul modo di realizzare una condizione di rispetto per la libertà e la dignità dei lavoratori. «Gli interessi dei lavoratori» - osservava Giugni - «saranno tutelati solo sulla base di una attiva iniziativa sindacale; una reale democrazia industriale si fonda infatti su un equilibrio di poteri tra rappresentanza dei lavoratori e direzione dell'impresa in un clima di libertà e legalità». È interessante notare come, al contrario di quanto sostengono oggi certe vulgate, la tesi portata avanti da Giugni, e che costituirà la base dello Statuto dei lavoratori, si rifacesse ad esperienze inglesi e soprattutto americane. In particolare, di quei Paesi si sottolineava l'apprezzamento positivo dell'organizzazione sindacale con base nella sezione d'azienda (il *local*) e si suggeriva implicitamente l'adozione di leggi che, come il *Wagner* *Act* americano, imponessero all'imprenditore il riconoscimento del sindacato ed un continuo dialogo con esso. La teoria di Giugni, che divenne patrimonio comune di un gruppo di studiosi diversamente orientati sul piano ideologico ma tutti definibili riformisti, proponeva in sostanza l'adozione di una normativa che, oltre a rimuovere gli ostacoli alla libertà di associazione nell'impresa, fosse promozionale o incentivante, e cioè attribuisse alle strutture aziendali del sindacato un ampio spazio operativo e alcuni fondamentali poteri. Verso la metà degli anni Sessanta, queste teorie finirono per imporsi almeno in parte del sindacato e a trovare interlocutori sempre più attenti nei settori culturalmente più aperti e moderni, anche se minoritari, della DC e del PSI. Come nota ancora Mancini, «si avverò, insomma, un fenomeno non troppo frequente nei rapporti tra giuristi e classe politica in Italia: quello di studiosi che, anziché agire da segretari del principe, e cioè mettere la loro tecnica al servizio delle forze istituzionali, operano come autentici specialisti della razionalizzazione sociale, elaborando una loro politica del diritto e favorendone l'accoglimento da parte di tali forze». L'emanazione di uno Statuto dei lavoratori comparve per la prima volta nelle linee programmatiche del primo Governo cosiddetto organico di centrosinistra, nel dicembre del 1963. Tuttavia, a parte l'approvazione della legge n. 604 del 1966 (un'altra tappa importante dei diritti dei lavoratori che non a caso oggi si cerca di colpire), si dovrà attendere la fine del 1968

Già vicesegretario della CGIL e successivamente del PSU, Brodolini fu il Ministro del lavoro al quale si devono, pur nel breve periodo del suo dicastero, una serie di riforme concrete in difesa dei diritti dei lavoratori quali il superamento delle gabbie salariali, la prima organica riforma previdenziale, provvedimenti di riforma del collocamento per abolire il sistema del caporalato, il risanamento del sistema mutualistico, oltre naturalmente al progetto dello Statuto, alla cui realizzazione dedicò tutte le sue forze e del quale tuttavia, a causa di una grave malattia, non riuscirà a vedere la realizzazione. Il progetto dello Statuto, elaborato nel 1969 dalla commissione tecnica del Ministero del lavoro presieduta da Gino Giugni, divenne il disegno di legge n. 738 dello stesso anno. Dopo un lungo e travagliato *iter* al Senato, dove il testo originale fu ampiamente emendato, venne approvato in tempi brevi alla Camera, dando vita alla legge 20 maggio 1970, Chiunque esamini senza pregiudizi il testo della legge non può non giungere alla conclusione che il baricentro positivo della disciplina sia individuabile nei Titoli II e III. Il Titolo II, di ispirazione chiaramente americana, assicura un ampio riconoscimento alla libertà di organizzazione e di azione sindacale (articolo 14) e la repressione delle pratiche sleali, ossia dei tipici comportamenti con cui l'imprenditore potrebbe vanificare l'esercizio di tale libertà. Mi riferisco agli articoli 15, 16, 17 e 18, ma anche al 22 e al 28. Il Titolo III costituisce il naturale sviluppo del precedente: una volta penetrata nell'impresa, la libertà sindacale non può esaurirsi nel riconoscimento del momento associativo, ma deve necessariamente espandersi fino a consentire l'attivazione di ulteriori strumenti in grado di dinamicizzare l'azione sindacale. Si attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali e se ne fa coincidere l'ambito con quello delle associazioni sindacali, così che possano prendere parte alla contrattazione

loro dirigenti è dato anche un modo di espletare le proprie funzioni mediante i permessi retribuiti e non retribuiti (articoli 23 e 24), l'attribuzione di un locale (articolo 27) e un'energica tutela contro il licenziamento e il trasferimento Oggetto di protezione e di promozione sono anche i sindacati in quanto tali. Ai sindacati esterni (soprattutto nei Titoli IV e V) e alle rappresentanze aziendali sono affidati compiti importantissimi, anche nel quadro della tutela specificamente rivolta ai lavoratori singoli. Un certo margine è lasciato anche ad altre possibili forme organizzative: l'articolo 14, oltre al diritto di associarsi, garantisce quello generico di svolgere attività sindacale; l'assemblea stessa può sempre esprimere una volontà autonoma dai sindacati (e ne abbiamo avuto esempi in anni recenti). La legge n. 300 del 1970, approvata nel mezzo del più intenso ciclo di lotte operaie verificatosi nella nostra storia (il biennio 1968-1970), mirava dunque a rafforzare, in un delicato equilibrio, la presenza del sindacato, sia nei confronti della controparte imprenditoriale sia nei confronti di una pressione da parte della base che potrebbe sfuggire al controllo delle organizzazioni. Certamente importante è l'idea di fondo, che riprende l'ispirazione fondamentale della Costituzione, di valorizzare il sindacato come agente di trasformazione sociale e di eguaglianza sostanziale. Un sindacato necessariamente forte, unito e intercategoriale in cui la compresenza, all'interno della stessa organizzazione, di diverse categorie costringe l'organizzazione stessa a coltivare e a trovare una sintesi tra le diverse esigenze, più facilmente al riparo dunque da visioni corporative. Assai diversa purtroppo è la situazione attuale. Il panorama sindacale oggi è caratterizzato da divisioni profonde e talvolta laceranti. È tuttavia sotto gli occhi di tutti come tale situazione, in un momento di crisi come quello attuale, anziché preoccupare venga sfruttata e spesso alimentata ad arte da quelle forze, sia politiche che economiche, che puntano al più classico *divide et impera*. Non si può negare che lo Statuto sia una legge "matura". Era ispirata ad una realtà industriale che oggi non esiste quasi più, in cui il modello di riferimento era costituito dalla fabbrica con migliaia di addetti, in maggioranza operai. Si trattava di una realtà in cui la modernizzazione delle relazioni industriali era non solo più necessaria ma anche, probabilmente, più facilmente praticabile. La realtà di oggi è innegabilmente assai diversa, caratterizzata in larga parte da piccole unità produttive e da un'espansione del terziario impensabile quarant'anni fa. È necessario tuttavia essere chiari. Se pure può essere riconosciuta la necessità di qualche eventuale correzione alla normativa dello Statuto, non possono esserne messi in discussione quei principi di fondo la cui validità non è stata mai messa in dubbio nemmeno dai critici più severi, ma intellettualmente onesti, della legge n. 300 del 1970. Sono a tal proposito da respingere con nettezza le pelose offerte di dialogo di certi settori politici che, dietro a formali dichiarazioni di intenti circa una semplice presunta volontà di modernizzazione del nostro diritto del lavoro, nascondono soltanto un ideologico desiderio di rivalsa antisindacale. A tal proposito credo che non ci siano parole migliori di quelle di quel Gino Giugni che dello Statuto fu il padre. Diceva infatti: «Sono trascorsi 35 anni e oggi nessuno metterebbe più in discussione l'idea di base dello Statuto, anche se qualche tentativo aleggia nell'aria. Mi riferisco soprattutto alle polemiche esplose in questi ultimi anni intorno all'articolo 18. (...) È vero, qualche anno fa prospettai la possibilità di un cambiamento dello Statuto, senza che questo volesse in alcun modo significare la cancellazione dell'articolo 18. Non era la prima volta che avviavo una riflessione sul tema. (...) Ma il fatto che io avessi lavorato con entusiasmo all'elaborazione dello Statuto, che mai ho smesso di difendere, non m'impediva di capire che il contesto che aveva prodotto quel complesso di norme era mutato. Oggi, tuttavia, sono convinto che i problemi del mondo del lavoro siano ben altri e che debbano essere risolti prima di mettere le mani sullo Statuto. Qualsiasi modifica in questa fase risulterebbe molto impegnativa e, inoltre, sarebbe necessario coordinarla con una ben ponderata riforma degli ammortizzatori sociali che, invece, non sembra essere una vera priorità per il mondo politico». Non possiamo, signora Presidente, che essere d'accordo.

lo Statuto dei lavoratori è stato approvato dal Parlamento italiano con la legge 20 maggio 1970, n. 300, esattamente 40 anni fa. Con tale documento sono stati regolamentati e tutelati i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti, inclusa la libertà del lavoratore dal punto di vista sindacale. La legge era nata in un clima di forte mobilitazione e di richiesta di cambiamento che non riguardava solo i lavoratori italiani, ma era diffuso in mezzo mondo. Nel nostro Paese il conflitto politico-sindacale raggiunge il culmine nel biennio 1968-69: periodo di acerrime lotte sindacali, duri scontri di piazza, occupazioni delle fabbriche. Non dimentichiamolo. Proprio in quel periodo, l'allora ministro del lavoro, Giacomo Brodolini, istituì una commissione nazionale per redigere una bozza di statuto, alla cui presidenza nominò appunto Gino Giugni, che ha anche steso il testo della legge, motivo per il quale gli è stato dato l'appellativo di «padre dello Statuto». Ma non dimentichiamo anche che la legge venne approvata in uno scenario in cui la tipologia contrattuale prevalente era il contratto di lavoro dipendente ed in cui parole come flessibilità, globalizzazione, delocalizzazione erano sconosciute al vocabolario del mercato del lavoro. E non scordiamo che la legge fu approvata con l'astensione del Partito Comunista, guarda caso quello stesso schieramento politico che oggi difende lo Statuto a spada tratta, accusando chi lo vuole riformare di voler ledere gli interessi ed i diritti dei lavoratori. Oggi quello Statuto compie 40 anni. E nel suo 40° anniversario anche noi della Lega riconosciamo che esso ha introdotto regole di civiltà, per cui i suoi principi vanno salvaguardati e - a mio parere - devono essere ritenuti intangibili. Ma è pur vero che in quarant'anni che in quarant'anni è mutato il contesto socio-economico, è cambiato il rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Pertanto, noi legislatori abbiamo il dovere di riformare, per adeguare la normativa alla realtà che cambia. Lo stesso Gino Giugni aveva riconosciuto l'opportunità di aggiornare lo Statuto in alcune parti. Ma in tema di riforme il mio pensiero va anche a Marco Biagi, che credeva fermamente nel processo di riforma. Voglio a tal proposito ricordare le sue parole: «Riformare il mercato del lavoro è la condizione per conseguire l'obiettivo di aumentare l'occupazione, accrescendone la qualità». Ed infatti le molte figure contrattuali introdotte dalla legge Biagi si sono tradotte in un aumento dell'occupazione. Delle sue idee molto è stato fatto, ma molto ancora resta da fare. La Lega Nord è per le riforme e crede in esse, per uno Stato progredito e competitivo, al passo con i tempi. Crediamo, dunque, sia giunto il momento di intervenire anche sulle tutele dei lavoratori, per estenderle ai lavori ed alle nuove forme contrattuali, tenendo conto dei diversi contesti produttivi, aziendali e territoriali.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, è la sera del Capodanno del 1968, la televisione trasmette un servizio in cui si racconta che il Ministro del lavoro, il socialista Giacomo Brodolini, fino a qualche anno prima vice segretario della CGIL, ha trascorso la notte con i lavoratori della fabbrica romana Apollon. Qualche settimana dopo Brodolini si reca ad Avola a ricordare due braccianti uccisi negli scontri con le forze dell'ordine, e lancia la proposta di Statuto. Brodolini, socialista ed espressione, insieme a Lombardi e Giolitti, della punta più avanzata del primo centrosinistra, volle far approvare il prima possibile lo Statuto dei lavoratori. Aveva chiamato accanto a sé alcuni studiosi, tra i quali Gino Giugni, che ebbe il compito di coordinare il lavoro che portò all'approvazione dello Statuto. Il Consiglio dei ministri, il 24 giugno 1969, presentò al Senato il testo dello Statuto. Appena venti giorni dopo, in una clinica svizzera, Brodolini moriva di cancro. I familiari diranno che non aveva mai voluto parlarne. È giusto ricordare, a quarant'anni dallo Statuto, quel Ministro che lo volle tenacemente. Una ricerca politica che veniva da lontano, fin dal 1952, quando Di Vittorio, al congresso di Napoli della CGIL, propose uno Statuto dei diritti dei lavoratori, riassunto nello slogan «la Costituzione nelle fabbriche», e diceva in quel congresso: «Il lavoratore è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa e vuole che questi diritti siano rispettati da tutti». Al nome di Di Vittorio e a quel lavoro Brodolini rimase per sempre legato. E lo Statuto è il coronamento del sogno di quel Ministro. L'*iter* parlamentare dello Statuto durò quasi un anno, fu coordinato da Gino Giugni ed ebbe il contributo di insigni giuristi tra i quali Federico Mancini, in particolare per l'articolo 18, e di un ex sindacalista, poi Ministro, che lo concluse, Carlo Donat- Cattin, cui si deve attribuire l'importantissimo articolo 28. L'opposizione contribuì a migliorare e correggere il testo, anche se poi, al termine del suo *iter*, decise di astenersi. La motivazione addotta per l'astensione, «la mancata adozione di un qualche *status* a favore dei partiti nel dibattito interno ai luoghi di lavoro», ancora oggi non mi appare convincente. Viceversa, mi ritrovo di più con l'interpretazione che nel 2006 diede Bruno lo Statuto dei diritti del lavoro (...) nel 1970 dava corpo alla grande idea di Di Vittorio di vent'anni prima. Purtroppo una parte della sinistra, i parlamentari del PCI, si astennero al momento della sua approvazione, solo perché» in quel momento «esclusa dalla Il lavoro di Brodolini e Giugni, portato a termine con il ministro Donat-Cattin, rimane una parte non cancellabile, per il suo portato di civiltà e di dignità del mondo del lavoro, del passato e del presente ma anche del futuro di questo Paese. A quant'anni dall'approvazione della legge 20 maggio 1970 n. 300, non possiamo non evidenziare come questa normativa sia a tutt'oggi un punto avanzato del nostro ordinamento giuridico. Normativa capace di attribuire ai lavoratori una dote di diritti di carattere universale tesi a declinare i valori della Carta costituzionale in diritti effettivi. Un complesso di garanzie che aveva ed l'ambizione di non incidere solamente nelle relazioni industriali, ma che attribuiva al lavoratore una dose importante di diritti di cittadinanza, attribuendo ad esso, attraverso lo strumento normativo, la tutela della libertà e della dignità del lavoratore, nonché il fattivo diritto di associazione sindacale nei luoghi di lavoro. Una dose di diritti, quindi, inalienabili ed universalistici, che non possono non essere attribuiti (anche se con diverse modalità) anche alle nuove forme di lavoro flessibili che si sono venute a determinare negli ultimi anni e che all'epoca dell'approvazione dello Statuto erano sostanzialmente inesistenti. Una legge moderna, ancora oggi attuale, ma spesso non applicata nel suo complesso. Una normativa che non ha attenuato il conflitto nelle relazioni industriali, ma che ha avuto il merito di ricondurlo entro un recinto di regole condivise. Una legge che più volte è stata sottoposta ad attacchi, per lo più di carattere politico, e che però in sua difesa ha visto, anche pochi anni or sono, un forte movimento popolare manifestare. A mio avviso, uno dei punti critici che ha impedito in quarant'anni la piena attuazione della legge e del suo portato culturale e politico è da ricercarsi nella mancata approvazione di una normativa organica sulla rappresentanza e la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro, normativa che viceversa vide la luce per il settore pubblico anche grazie al prezioso lavoro di Massimo D'Antona, dal barbaro assassinio del quale proprio In conclusione, a quarant'anni dall'approvazione dello Statuto, voglio ricordare le parole di Umberto Romagnoli, uno dei grandi maestri del diritto del lavoro: «Il lavoro è senza aggettivi, non c'è lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, c'è il lavoro che è il passaporto della cittadinanza, come intende l'articolo 1 della Costituzione. Poi, il lavoro non deve essere solo l'oggetto di un contratto, ma il modo attraverso cui la cittadinanza esiste, ha una sua visibilità, reclama una presenza e uno spazio. Per cui se fino ad ora i sindacati hanno rappresentato e tutelato il cittadino come lavoratore, adesso devono imparare a rappresentarlo in quanto cittadino». Nel momento in cui, insieme, ricordiamo i quarant'anni dello Statuto, non possiamo però dimenticare i troppi progetti di legge che ne stravolgono i contenuti. Noi Democratici a quei principi della legge n. 300 siamo e resteremo fedeli.

Presidente, colleghi, la capacità di dialogo tra maggioranza e opposizione, insieme all'esigenza di adeguare il nostro sistema giuridico alla nuova realtà economica e sociale, portarono nel '70 all'approvazione della legge n. Oggi, a quarant'anni di distanza, lo Statuto dei lavoratori continua a far discutere e a dividere tra coloro che lo considerano una conquista di civiltà e coloro che vorrebbero cambiarlo. Con esso, ci si poneva l'obiettivo di istituire e regolare il rapporto di lavoro inteso come rapporto sociale e non come rapporto di mercato. Si stabiliva una regola sociale: «uno strumento per cambiare il potere dentro la fabbrica e una prefigurazione normativa del mondo operaio di partecipare al governo dell'impresa». L'identità personale del lavoratore finiva per coincidere con quella identità collettivo-sindacale. Proprio per questo lo Statuto garantisce in modo particolare la libertà sindacale e promuove l'autonoma organizzazione sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La teorizzazione di una legislazione di sostegno o promozionale mirava poi - per usare le parole di Giugni ad incoraggiare e garantire la contrattazione e gli autori di essa, rimuovendo gli ostacoli giuridici e di fatto, ponendo in essere più avanzate condizioni legali e di esercizio che non fossero quelle di mero diritto comune. Lo Statuto dei lavoratori con la sua architettura complessa è stato capace di armonizzare, sotto l'impulso innovatore di Giacomo Brodolini e Gino Giugni, due differenti ispirazioni: quella di assicurare al sindacato la piena cittadinanza all'interno delle fabbriche e quella di permettere al lavoratore l'esercizio dei diritti consacrati dalla Carta costituzionale. Seguendo la prima ispirazione, ad una visione paternalistica del rapporto di lavoro, che vedeva il lavoratore come soggetto debole sottoposto al potere e all'autorità del datore, il legislatore sostituisce un modello di gestione dei rapporti di lavoro costruito attorno alla tutela della «libertà e della dignità del lavoratore». La seconda ispirazione si sintetizza emblematicamente nello slogan «la Costituzione nelle fabbriche». Caduto il sistema corporativo del ventennio, due principi della Costituzione hanno retto per lungo tempo l'insieme dei rapporti intersindacali in Italia: l'articolo 39, secondo cui «l'organizzazione sindacale è libera», e l'articolo 40, secondo il quale «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Troppo poco perché l'azione sindacale trovasse spazio nella realtà quotidiana del mondo del lavoro, almeno fino a quando la stagione del '68 non riaprì la questione sociale riproponendo il tema della democrazia sindacale. Con la legge n. 300 si intese tradurre, sul piano della concretezza dell'agire quotidiano, i principi enunciati dalla Costituzione. Lo Statuto affonda infatti le sue radici negli stessi capisaldi che si ritrovano negli articoli 2 e 3 della Costituzione, recitano: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità»; personalità»; «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Altro principio costituzionale che ha ispirato lo Statuto è quello per il quale, dopo aver riconosciuto la libertà di iniziativa economica privata, si afferma che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana» A questi e ad altri principi costituzionali rinviano quelle norme dello Statuto dei lavoratori che garantiscono la libertà di opinione nei luoghi di lavoro (articolo 1), vietano l'effettuazione di indagini sulle opinioni politiche, religiose gli atti discriminatori posti in essere per motivi sindacali, politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso (articolo 15), o ancora i divieti di sindacati di comodo Già trattando di questi istituti, ma anche a proposito dell'effettività del contraddittorio in tema di sanzioni disciplinari (articolo 7), della tutela della salute e dell'integrità fisica, che i lavoratori possono condurre mediante loro rappresentante la presenza del sindacato. Questa viene organicamente sistematizzata, secondo l'articolo 14, con la garanzia, assicurata «a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro», di poter «costituire associazioni sindacali, aderirvi e svolgere attività sindacale». Viene, inoltre, meglio specificata dall'articolo 19 che prevede che in ogni unità produttiva possano essere costituite rappresentanze sindacali aziendali l'architrave, la chiave di volta dell'intero edificio non può non essere ravvisata negli articoli 18 e 28, ovvero nell'istituto della reintegra nel posto di lavoro e nelle procedure di repressine della condotta antisindacale. A dimostrazione del valore intrinseco e delle capacità espansive dei principi contenuti nello Statuto sta l'accoglimento di molti di essi nello stesso testo della cosiddetta Carta di Nizza: mi riferisco agli articolati divieti di discriminazione, ai diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, fino al diritto di negoziazione e di azioni collettive con particolare riguardo alla «tutela contro ogni licenziamento ingiustificato». All'epoca della sua promulgazione lo Statuto dei lavoratori fu fin da subito definito come elemento innovativo, in grado di chiudere un periodo di evoluzione sociale del tessuto produttivo italiano stabilendo una mediazione tra capitale e lavoro. Da alcuni fu criticato per la sua timidezza, da altri per la sua eccessiva incisività. Tutte le critiche e gli elogi al legislatore avevano in comune il riconoscere che si trattava comunque di una norma in grado di regolamentare un equilibrio sociale dentro le fabbriche, in cui il capitale poteva mantenere le proprie prerogative in una fase di espansione del conflitto sociale, dovendo però riconoscere al lavoro una sua dignità, alla forme collettive di associazione dei lavoratori un ruolo nella vita aziendale. Ora, viene spontaneo chiedersi: a 40 anni dal suo varo, è ancora attuale? Ovvero, mutato il contesto, si deve determinare necessariamente un mutamento del prodotto giuridico? Il giudizio storico su questa legge non può che essere positivo: i protagonisti della vicenda hanno dimostrato una capacità di leggere i cambiamenti della struttura economica e sociale della nostra società e di avanzare proposte adeguate che non si limitavano alla situazione contingente. I conflitti c'erano ed erano aspri, eppure gli attori, individuali e collettivi, furono in grado di collocare gli interessi che rappresentavano in un ampio e significativo orizzonte assumendo, come tavola di valori condivisi, la Costituzione, che consentì sia il dialogo che compromessi ragionevoli. Tuttavia, lo Statuto è una legge che va applicata ancora oggi ed è dunque necessario riflettere sull'attualità dei suoi contenuti normativi. Lo Statuto venne approvato, ma il capitalismo industriale cominciò da quel momento a cambiare pelle, con le esternalizzazioni e il decentramento produttivo. Le imprese si alleggerirono e lo Statuto, che aveva come modello di riferimento la grande impresa fordista, verticalizzata, venne svuotato progressivamente da questo processo. L'assetto delle relazioni industriali e sindacali che ha prodotto lo Statuto non c'è più, parte dei suoi contenuti normativi tuttavia sono ancora attuali: le norme a tutela della libertà e dignità del lavoratore, le norme di sostegno all'attività sindacale nei luoghi di lavoro, le norme di attuazione, per quanto riguarda il lavoro, della Costituzione, patto fondamentale della nostra convivenza. Tuttavia, oggi, di fronte alla separazione del lavoro dall'impresa, alla centralità della segmentazione del processo produttivo, all'esternalizzazione, alla disomogeneità e disaggregazione della forza lavoro, non possiamo sottrarci ad una riflessione sulle urgenti esigenze di aggiornamento e di modifica dello stesso e sul suo adeguamento all'attuale contesto. Siamo consapevoli del fatto che lo Statuto dei lavoratori abbia un forte valore simbolico oltre che normativo. Per questo, riteniamo che ogni necessario e opportuno cambiamento o ammodernamento dovrà ispirarsi ai principi che ne furono il fondamento: i rapporti di produzione sono subordinati ai valori costituzionali, il lavoro non è una merce, deve essere promozione della persona umana e partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lo sforzo della politica oggi dovrebbe essere quello di dar vita a una vera "Costituente sociale", che si faccia carico dell'individuazione ed attuazione di nuovi principi di equità, fra lavoratori e fra territori del territorio nazionale. In tal senso, dare attuazione all'articolo 39, evitare le riaffioranti suggestioni delle gabbie salariali, impedire - come giustamente sostiene presidente Fini - che la flessibilità equivalga alla precarietà, rendere più responsabili i lavoratori, regolamentando la loro partecipazione alla vita e agli eventuali utili dell'azienda, sono impegni che non solo il Governo ma tutte le forze politiche e le parti sociali devono assumere per rendere effettivo il diritto al lavoro e il dovere di lavorare bene. Con queste parole e con lo sguardo al futuro, rivolgiamo ai lavoratori, al purtroppo vasto mondo del precariato, ai disoccupati italiani, e in particolare a quelli del Mezzogiorno, l'augurio che la saggezza politica prevalga e che negli anni a venire, piuttosto che parlare di tagli agli stipendi, si possano realmente offrire occasioni di lavoro, di lavoro vero e di lavoro duraturo.

questo Statuto. Nella mia memoria è ancora presente il ministro Brodolini che, con la sciarpa bianca, una notte fece alcune dichiarazioni molto importanti relative al mondo del lavoro. Io ricordo con simpatia

300 del 1970, di cui parliamo oggi, credo sia la fonte normativa più importante. Qualcuno l'ha definita la Costituzione in materia di libertà ed attività sindacale. Ed è un esempio: oggi ci deve essere di esempio di unità,

e cambiò radicalmente, a mio parere, le condizioni in fabbrica dei lavoratori; si determinò una rivoluzione culturale e politica con l'approvazione di questa legge. Purtroppo oggi, signor Ministro, è un anniversario triste

Ecco perché bisogna utilizzare questo anniversario per una seria riflessione, che certamente non può che riaffermare il valore dei principi, soprattutto di quelli contenuti nel Titolo I della legge. 300.

di questa importante legge. La prima parte della legge costituisce ancora la piattaforma fondamentale dei diritti civili e sociali della persona umana. Per questo non siamo entusiasti di passare, come qualcuno oggi ha detto, dallo Statuto dei lavoratori allo Statuto del lavoro. Riconfermiamo la validità di fronte al lavoro della persona umana, la centralità della persona umana, di cui siamo portatori in politica ed anche nella società.

però con atteggiamento punitivo, come sembra emergere da alcune dichiarazioni, ma consapevoli che dobbiamo scrivere maggiori tutele per i lavoratori, soprattutto, come ricordava qualcuno, per la moltitudine di lavoratori atipici, che certamente nel '70 non si conoscevano (precari, lavoro esternalizzato e così via). Questo è il vero dramma che la politica di oggi deve assolutamente risolvere. Si tratta di riscrivere una moderna Carta dei diritti e delle tutele, che non trascuri le diversità esistenti nel mondo del lavoro, ma che articoli le strategie di tutela e di valorizzazione delle persone in rapporto ai diversi ambiti e modalità in cui si esplica la loro attività lavorativa. Bisogna garantire il diritto del lavoro come inderogabile per tutti e la contrattazione collettiva di massa; sostenere, sì, la mobilità del lavoro - nessuno vuole essere retrogrado o non abbracciare le nuove forme di lavoro - ma accompagnata da una formazione professionale mirata: per esempio, perché non parlare di un salario minimo garantito nel nuovo Statuto dei lavoratori?. Occorre fissare i diritti dei cittadini anche all'esterno della fabbrica e del mondo del lavoro (per esempio, il reddito sociale minimo). Si presenta l'occasione per poterne discutere e per dare questi diritti ai giovani di oggi che vanno alla ricerca del lavoro.

dividere le forze sindacali. Proprio in questi giorni ne abbiamo un esempio. Oggi ci auguriamo anche che si realizzi la partecipazione del lavoratore all'impresa - l'altro capitolo

i punti fondamentali del nuovo Statuto. Auguriamoci che questa giornata serva a rivitalizzare il dibattito e a ricostruire un nuovo sistema di protezioni. Nel 1970 intervenne un accordo generale: oggi va ricreato lo stesso clima di collaborazione, per potere riscrivere parte dello Statuto, nel rispetto del lavoro e dei lavoratori. le iniziative di questo Governo in materia non mi piacciono, ed alimentano diffidenze e preoccupazioni. Il lavoro e i lavoratori meritano più rispetto ed unità.

Basta fermarsi a pensare alle condizioni del mondo del lavoro dipendente e delle relazioni sindacali nel 1970 ed a quanti cambiamenti sono intervenuti nel mercato del lavoro. 300 del 1970 venne approvata nel mezzo del più intenso ciclo di lotte operaie della nostra storia e mirò a rafforzare la presenza del sindacato, sia nei confronti della controparte imprenditoriale, sia nei confronti di una base sempre più difficile da controllare. La legge, evidentemente pensata e scritta per la realtà industriale della fabbrica, risultò scarsamente incisiva sulle piccole unità produttive. Inoltre, il rapporto di lavoro era tendenzialmente "per sempre": avere un posto sicuro, fisso, era non solo un obiettivo, ma la normalità. Chi entrava in un'azienda lo faceva con la consapevolezza che, a meno di eventi straordinari o di scelte individuali, avrebbe trascorso in quell'ambiente l'intera sua vita lavorativa fino al momento del collocamento a riposo. Nel 1970 non esistevano i lavoratori a progetto, né quelli a chiamata: o ci si metteva in proprio o si era dipendenti. Conseguentemente, la legislazione legislazione posta a tutela dei dipendenti era tesa al mantenimento del posto fisso e al miglioramento delle condizioni di vita aziendale. Già solo queste brevi considerazioni iniziali fanno sì che appaia subito evidente quanto la legge n. 300 del 1970 sia uno strumento purtroppo inadeguato a realizzare la tutela di tutte quelle figure e fattispecie lavorative via via introdotte e modificatesi nel corso degli anni. Per quanto riguarda la parte rivolta ai diritti sindacali, è sotto gli occhi di tutti quanto il mondo della rappresentanza si sia evoluto negli ultimi decenni. È all'incirca dalla metà degli anni Ottanta che il sindacalismo confederale, pur tendenzialmente egemone grazie ad un sistema di regole che gli consente di autotutelarsi, registra una grave crisi di rappresentatività, cioè una perdita della capacità di esprimere in modo credibile gli interessi di un ampio spettro di lavoratori. Molteplici ne sono le cause, e possono distinguersi in strutturali e funzionali. Tra le prime, vanno annoverate la rivoluzione tecnologica, la crescente terziarizzazione dell'economia, l'accesa competitività internazionale: queste, importando una profonda trasformazione delle tecniche di produzione e di organizzazione del lavoro, hanno favorito il mutamento del corpo sociale e la sua diversificazione, con l'emersione di nuove professionalità e nuovi mestieri e l'esplosione del lavoro parasubordinato. Di qui la tendenza alla desindacalizzazione e alla frammentazione del panorama sindacale. I lavoratori non sono più monopolio di poche grandi organizzazioni sindacali (che anzi hanno perso e continuano a perdere consenso), ma si sono organizzati sempre più in sindacati di categoria, di base e soprattutto in sindacati territoriali, capaci di essere più vicini, più sensibili ai problemi di chi quotidianamente deve far quadrare i conti della spesa e confrontarsi con l'inadeguatezza dei servizi alla persona e alla famiglia. Tra le seconde cause va annoverato, invece, il passaggio ad una contrattazione "in perdita", cioè distributiva di sacrifici. In poche parole, il vecchio sindacato è visto dai lavoratori più attento a preservare i propri diritti e privilegi, piuttosto che a impegnarsi per ottenere una ripartizione equa dei sacrifici e nella tutela delle nuove figure maggiormente professionalizzate rispetto alla massa operaia tipica delle aziende degli anni Settanta. Alla luce di questi cambiamenti, è nella logica delle cose che non sia più rinviabile una riforma del diritto sindacale che garantisca ai lavoratori la possibilità di scegliere da chi farsi rappresentare ed alle organizzazioni che li rappresentano la possibilità di poter contare su strumenti legislativi moderni che consentano loro di svolgere la propria attività di contrattazione e di tutela dei propri iscritti in virtù del consenso nelle aziende, e non di un'autoreferenzialità che ricorda il diritto divino dei monarchi assoluti. Lo Statuto aveva quindi fotografato la realtà dell'epoca e aveva cercato di dare la miglior risposta possibile alle esigenze dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Ma, si sa, le leggi non sono altro che forme d'ordinamento di processi sociali che si sono ormai assestati e consolidati. Nello scenario odierno, questa legge è evidentemente segnata dai limiti ideologici di un'epoca ormai trascorsa e lontana: la centralità egemonica della classe operaia della grande impresa, l'inamovibilità dal posto di lavoro, occupato dall'apprendistato alla pensione. Ogni strumento vale solo fino a quando è utile: quando diventa inadeguato rispetto ai tempi e ai cambiamenti bisogna avere il coraggio di metterci mano. Per queste considerazioni siamo profondamente convinti che l'attuale Statuto dei lavoratori debba essere sostituito da uno strumento più moderno, che sappia tutelare anche le nuove forme di lavoro subordinato e parasubordinato e consentire ai lavoratori di organizzarsi sindacalmente nelle forme che che più preferiscono, eliminando corsie preferenziali (si pensi ai limiti del ricorso all'articolo 28, nei fatti appannaggio di poche organizzazioni), nella direzione di garantire finalmente una vera pluralità e la democrazia sindacale.

ma, a maggior ragione, se l'apprezzamento riguarda il passato poi deve tradursi in significati politici per il futuro. Una prima osservazione, se vogliamo fare un'analisi lucida e, se volete, anche aiutata dalla distanza, dovrebbe distinguere il significato e i principi dello Statuto dalle singole norme Molte di queste sono invecchiate, altre sono state cambiate: quindi, lo Statuto non è più quello di un tempo, ma in realtà i princìpi che lo sostanziano sostanziano sono di rango costituzionale e, giustamente, poi sono stati riprodotti ed allargati a livello internazionale e, di recente, nella Costituzione europea, il che è bene ricordare anche qui. Questi principi sono ancora la piattaforma dei diritti fondamentali civili e sociali della persona che, allora, lo Statuto fece entrare nei cancelli della fabbrica.

Questa parte dello Statuto, soprattutto la prima, è servita a costituzionalizzare il potere dell'imprenditore di allora e ha una funzione tuttora attuale, se non altro perché costituisce una remora a possibili involuzioni della prassi di gestione del personale. In un momento così difficile, questa non è una funzione da poco.

ha garantito il pluralismo e l'autonomia del sindacato, nonostante non sia stata poi integrata, come invece avrebbero voluto Giugni e gli autori di allora, da una pratica

Queste sono le due grandi indicazioni che ci vengono da allora. Detto questo, guardando avanti, bisogna riconoscere che ci sono dei punti critici. I diritti individuali e collettivi che allora furono sanciti, e che valgono anche adesso, hanno ridotto, ma non cancellato, l'asimmetria di potere che caratterizza i rapporti di lavoro. È bene dirlo, perché qualcuno sembra pensare che non sia più così. Soprattutto, questo è il problema maggiore, la normativa di allora è diventata incompleta e insufficiente - com'è stato ricordato - per per fronteggiare le nuove realtà del mondo del lavoro, in particolare la diversificazione dei lavori, dai precari agli atipici, ma anche

tecnica, ma con un'ispirazione di base che resta. Infatti, l'idea di base dello Statuto, quella dei diritti fondamentali individuali e collettivi, è tanto presente oggi - noi lo vogliamo sottolineare - che anche quando si ricercano forme di regolazione dei nuovi lavori, si usa la parola «statuto». Io vorrei mantenerla, anche se magari lasciando perdere lo Statuto dei lavori. In sostanza, la sfida di oggi è applicare quell'idea di diritti fondamentali in un contesto molto più diversificato e più complicato, che quindi non abbia paura delle diversità esistenti nel mondo del lavoro, ma articoli le tutele e anche gli interventi di promozione - non si tratta infatti solo di tutelare il lavoro, ma anche di promuoverlo - in rapporto alle diverse modalità con cui il lavoro si manifesta. Se non lo facessimo, tradiremmo lo stesso obiettivo dello Statuto, che era appunto quello di sostenere e promuovere il lavoro secondo le proprie

delle condizioni di lavoro attuali, una base sociale comune e poi una diversificazione a seconda delle condizioni, perché questa è la sfida. Allora, lo Statuto ricompose, favorì le condizioni di lavoro in una fabbrica fordista accomunata Questa è la prima e più importante sfida che ci aspetta, e che lo Statuto può sostenere, ma va poi ma va poi affrontata con lo stesso spirito riformista e riformatore di allora. Il ripensamento riguarda i diritti e le tutele individuali dei diversi lavori, ma anche i rapporti collettivi, anche se se ne parla meno.

bisogna perseguire lo stesso obiettivo di bilanciamento dei poteri - Gino Giugni ricordava sempre: *checks and balances* - anche al di fuori della fabbrica, perché le decisioni imprenditoriali che influiscono sul lavoro sono sempre più spesso attuate anche al di fuori dell'impresa. Quindi, se vogliamo essere effettivi - come deve essere il lavoro - dobbiamo allargare l'orizzonte appunto al di fuori della fabbrica, ai rapporti che intervengono sul mercato del lavoro con le istituzioni e con le parti sociali, che sono sfidate molto più direttamente dalla legge. Questi sono due aspetti su cui lo spirito dello Statuto deve essere ripreso, anche per alimentare la ricerca di soluzioni nuove.

lì e che ci auguriamo vengano esaminati, perché ormai la protezione del valore del lavoro, in un contesto così mutevole, non si può più affidare solo a tutele normative, ma abbisogna di procedure di partecipazione e di controllo

intervento è dedicato soltanto a sottolineare un aspetto della vicenda dello Statuto dei lavoratori del 1970 che è stato forse tenuto indebitamente in ombra nel dibattito di questi giorni. L'elaborazione e l'emanazione dello Statuto hanno coinciso con la crisi di una corrente di pensiero molto importante, quella che va sotto il nome di «contrattualismo sindacale» e che ha caratterizzato particolarmente l'elaborazione teorica ed il comportamento pratico di una grande confederazione sindacale italiana, la CISL. Lo Statuto ha avuto il merito di recepire e generalizzare i contenuti fortemente innovativi della contrattazione collettiva della seconda metà degli anni '60 e, in particolare, dell'autunno caldo del '69. La sua emanazione, tuttavia, ha segnato uno spartiacque tra una legislazione in materia di lavoro rispettosa del principio contrattualistico e del principio di sussidiarietà, ed una legislazione, invece, fortemente invasiva, intrusiva ed ipertrofica, quella che ha portato la raccolta delle leggi vigenti nel nostro Paese in questo campo ad occupare quasi 3.000 pagine, caratterizzate oltretutto da grave disorganicità, ma, soprattutto, da un grave difetto di effettività: alla dilatazione del volume normativo ha corrisposto una riduzione del campo di applicazione effettiva della legge. Lo Statuto - che pure nell'immediatezza della sua emanazione venne tacciato di essere una legge malfatta - è stato invece esemplare per semplicità, chiarezza ed aderenza agli equilibri del sistema di relazioni industriali. Subito distribuito in milioni di esemplari in ogni luogo di lavoro, in ogni angolo del Paese, esso in pochi mesi ha saputo cambiare profondamente la cultura del lavoro nel nostro Paese,

Questi beni inestimabili - semplicità, chiarezza, effettività, aderenza agli equilibri del sistema di relazioni industriali - sono però andati ben presto perduti nella nostra legislazione del lavoro. Nel momento in cui celebriamo i 40 anni di questa legge straordinaria, credo che dobbiamo assumere l'impegno, un impegno possibilmente *bipartisan*, a recuperare questi beni ed, in particolare, a ristabilire un corretto rapporto tra sistema delle relazioni industriali e legislazione del lavoro. Consapevoli che quando - come oggi diffusamente accade - la legge viene di fatto disapplicata, è la democrazia stessa ad essere messa fuori gioco.

credo davvero che il senso di questa celebrazione debba essere trovato nel proporre alcune riflessioni, magari eccentriche e non convenzionali, che però possano trasformarsi in materiale utile per un necessario intervento di compimento di quella traiettoria di modernizzazione che nello Statuto dei lavoratori trovò un momento autentico, dispiegato e fondante. La prima eccentricità - se mi è consentito - è quella rispetto alla *lectio facilior*, dominante anche nel dibattito degli ultimi giorni, in ordine alla filiazione diretta da parte dell'«autunno caldo», dello Statuto dei lavoratori. Come ogni *lectio facilior*, corre il rischio di essere assai seducente, ma anche molto sdrucciolevole.

tra l'orizzonte di senso, in termini di regolazione del mercato del lavoro e del diritto del lavoro, che ha trovato compimento nello Statuto, e invece quanto accadeva nelle proposizioni ideologiche dei movimenti. Basti pensare a chi furono davvero i protagonisti della manifattura dello Statuto dei lavoratori: Giacomo Brodolini, Gino Giugni il primo socialista a vocazione interna e il secondo socialista a vocazione internazionale - e Carlo Donat-Cattin. È dalla fusione feconda, vivace e propulsiva di quelle due culture, il socialismo riformista e il personalismo cattolico, che nasce la qualità più propria, più densa e più significativa della complessiva proposta dello Statuto dei lavoratori, che non a caso scandisce il quadro legislativo, ma immagina di dover riempire quel *frame* attraverso l'affidamento alle parti sociali di una dimensione propulsiva ed innovativa: ecco, dunque, la continuità della modernizzazione. Pare quasi di cogliere come, rispetto alla deriva sentimentale dei movimenti, lo Statuto dei lavoratori abbia rappresentato una sorta di ancoraggio razionale. Verrebbe la voglia, citando categorie elaborate in altro capitolo del diritto, di contrapporre un diritto del lavoro del *Gefuhl*, del sentimento, ad un diritto del lavoro del *Gesinnung*, cioè dell'atteggiamento interiore.

È evidente che, rispetto all'impostazione del Partito Comunista Italiano, lo Statuto dei lavoratori fu interpretato assecondandone la vocazione di senso attraverso la personalità dei suoi padri. suoi padri. A quella astensione, tra l'altro, seguì un dibattito molto acre nella stessa CGIL, la quale formulò una serie di proposizioni fortemente critiche. Questo sta a significare come in qualche modo lo Statuto dei lavoratori, con la sua razionalità e la sua vocazione contrattuale, si frapponesse al tentativo del Partito Comunista di allora di far dilagare nelle fabbriche la sua concezione antagonistica delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, fondata come tale, da un lato, sulla politicizzazione come vettore del conflitto sociale e, dall'altro, sul rifiuto dell'autonomia come elemento fondativo dell'azione sindacale. Non è un caso che si creò una complicità di fatto con pezzi dominanti della Confindustria di allora, che colsero nello Statuto dei lavoratori una minaccia all'esorbitare dell'unità degli approcci, che in qualche modo finirono per legittimare una prassi tutta difensiva rispetto all'applicazione dello Statuto. Due furono le conseguenze, certo segnate dell'eterogenesi dei fini, ma in qualche modo clamorose. Una fu lo scivolare della piccola impresa in un cono d'ombra irrimediabile. Per quasi sessant'anni la piccola impresa è stata condannata ad astenersi dal considerare le relazioni industriali come motore della propria propulsività economica, come vettore della propria capacità competitiva nell'arena internazionale. Si mescolarono poi due sindromi in qualche misura concorrenti. Da un lato, c'era la «sindrome del Lingotto», del Lingotto», che vedeva insieme la più grande impresa italiana, il più grande sindacato italiano e il più grande partito dell'opposizione italiana in una logica antagonistica nei presupposti e alla fine collusiva e consociativa nelle applicazioni quotidiane di un modello di relazioni industriali.

che il fascismo volle promuovere in luogo della vocazione autenticamente sussidiaria di quel corporativismo che era stato l'anima della dottrina sociale della Chiesa e delle fondative riflessioni sull'economia sociale di mercato negli anni '30. Quindi, questo condanna, attraverso la coazione, ad avere solo il contratto nazionale come punto di riferimento per le nostre piccole imprese, le quali si ritrovarono in un contesto nel quale, oltre il 50 per cento della catena del valore essendo valore del lavoro, esso fu affidato alla terzietà lontana, distante, incomprensibile, inapplicabile del contratto nazionale, comprimendo energia competitiva, denegando opportunità e traiettorie di sviluppo. L'altra sindrome è quella che in qualche modo condusse la grande impresa italiana a trascurare l'investimento valorizzante sulla risorsa umana come tracciato per lo sviluppo competitivo, preferendo quasi una sorta di insistita linea di investimento sempre e soltanto sul processo, sul prodotto, sull'impianto, sulla macchina nella sua funzione elusiva della risorsa umana, di quel sistema integrato di intelligenza, esperienza e competenza che è la risorsa umana che, culturalmente e antropologicamente connotata, genera prodotto. A questo - va detto con molta molta lealtà - ha dato un suo contributo anche un'applicazione per certi versi distorsiva dello Statuto dei lavoratori da parte della magistratura: magistratura italiana in qualche misura essa stessa permeata di spirito centralistico e burocratico, che ha sempre avuto una vera vocazione antisindacale nel nostro Paese. Un commentatore con simpatica acidità ebbe a dire che, se l'articolo 28 di quel medesimo Statuto dei lavoratori fosse stato applicabile alla magistratura, la magistratura stessa se ne sarebbe dovuta fare, di ordinanze contro se stessa, su quell'articolo! Noi tutti abbiamo memoria di un approccio dilatatamente intrusivo rispetto all'autonomia delle parti sociali e alla libera determinazione dei contenuti contrattuali da esse praticate. La magistratura portò sempre con sé l'idea di considerare lo Statuto quasi uno strumento per cancellare ogni possibilità di ricomposizione, di riconciliazione comunitaria nell'unità organica dell'impresa. Ci fu sempre l'idea di considerare lo strumento Statuto dei lavoratori per alterare

della Costituzione, partecipazione e sussidiarietà: cioè esattamente il contrario di quella che divenne in qualche modo, attraverso un percorso di eterogenesi dei fini, la condanna nella quale lo Statuto dei lavoratori si trovò proprio nel momento in cui, invece, completamente diverso era lo spirito informatore di coloro i quali lo avevano voluto.

grande paraclasi, di una grande faglia sociale; quando cioè da una parte ci sono gli *insider*, i garantiti, i protetti dalla munitissima cittadella dei diritti,

Credo che questa sia stata un'altra delle non volute condizioni a cui un'interpretazione male accorta dello Statuto ha portato, rispetto alle quali bisogna intervenire. l'appello che in qualche misura rivolgo al ministro Sacconi e, attraverso lui, al Governo è di intervenire prontamente per recuperare quella traiettoria di modernizzazione alimentata dalla tradizione che abbiamo individuato essere come il momento culturalmente propulsivo di un diritto del lavoro che sappia farsi accompagnatore vivace di una complessiva rinascenza dell'industria italiana, in due direzioni: la prima, secondo la profonda intuizione di Marco Biagi, cioè trasformando lo Statuto dei lavoratori in Statuto dei lavori. Il Ministro sa bene come questo lascito di Marco, contenuto nell'ultimo *file* al quale aveva lavorato la notte prima di essere assassinato e teneramente intitolato al nome della moglie Marina, sia la piattaforma dalla quale partire per realizzare quest'operazione, in cui si abbassano le mura della tutela di coloro i quali sono protetti dalla cittadella, ma si estende sino agli estremi confini del mondo in cui operano i protagonisti del lavoro e dell'impresa l'area di intervento, l'area di intervento, di agibilità, di praticabilità e di effettività delle tutele. Un *trade off* virtuoso, fatto magari di tutele leggermente più basse, ma infinitamente più estese, come capacità di presidio.

se il diritto del lavoro italiano è stato sempre segnato dall'affidamento della trazione alla legge, oggi è tempo che al contratto sia riconosciuto passare cioè da un modello "*push*", in cui la legge sostiene e invece spesso zavorra il crescere della società civile e delle dinamiche competitive, ad un modello "*pull*", nel quale invece è il contratto, è la rete delle determinazioni contrattuali delle parti nel concreto quotidiano della vita delle imprese che deve trascinare, attraverso le sue pratiche migliori, un generale sviluppo del Paese. Questo, signor Ministro, credo sia il modo migliore per celebrare lo Statuto dei lavoratori. So che lei nel pomeriggio intitolerà a Giacomo Brodolini e a Carlo Donat- Cattin alcune aule del suo Ministero che altre aule ha già intitolato a quel Massimo D'Antona, riformista vero, di cui ricorre oggi l'11º anniversario dell'assassinio, e a Marco Biagi. Ecco, in questo collegamento non banale, ma vero, autentico, commosso, alla storia di tutti coloro i quali hanno fatto della battaglia per la modernizzazione stia il modo più vero per riconoscere la tradizione di civiltà del nostro Paese: credo, signor Ministro, che in questo stia davvero

Signora Presidente, ringrazio tutti i colleghi intervenuti, soprattutto quelli di loro che hanno avuto la pazienza di ascoltarsi reciprocamente e, a questo punto, anche di ascoltare il rappresentante del Governo in un confronto che non è stato dedicato soltanto a celebrare - com'è doveroso

alla verifica circa l'attualità di quello Statuto e all'esigenza di eventuali integrazioni e correzioni, in modo che esso viva anche nella realtà che così straordinariamente cambia.

Anche quest'ultimo ricordo, e l'omaggio che rendiamo a Massimo D'Antona, dovrebbero indurre a riflettere circa i modi con i quali ci si deve confrontare sui

procedere ad ulteriori riforme in modo quanto più condiviso, perché le regole del lavoro appartengono in fondo alla Costituzione materiale del nostro Paese, che ovviamente si evolve e dovrebbe evolversi in termini largamente condivisi. Questo è stato anche il senso del modo con cui abbiamo prodotto il Libro bianco attraverso la pubblica consultazione, proprio nella convinzione che il futuro del modello sociale, che include la regolazione dei rapporti di lavoro, e lo sviluppo delle relazioni industriali che ne dovrebbe derivare costituiscano parte del nostro patto sociale. Osservo la necessità di un dibattito sereno, perché anche allora non ci fu soltanto un dissenso: se leggo la dichiarazione di voto dell'onorevole Giuseppe Sacchi, del Partito Comunista, non posso non fare una riflessione rispetto ad un atto poi così largamente condiviso. Anche allora, un legittimo dissenso, che va collocato nel contesto di quel tempo, ma si sottolinea tale dissenso con un linguaggio - e, a parte il linguaggio, con contenuti - di radicale contrapposizione. Disse l'onorevole Sacchi: «Se la maggioranza di questo Parlamento vorrà assumersi la responsabilità di approvare una legge che autorizza i padroni a continuare a calpestare la Costituzione nei luoghi di lavoro, ebbene di questo atto giudicheranno i lavoratori e non sarà certo un giudizio positivo per la maggioranza, ma una severa condanna». Oggi, per il solo fatto che io abbia ipotizzato l'evoluzione dello Statuto dei lavoratori verso lo Statuto dei lavori, ex parlamentare della sinistra dice: «Sacconi vuole i lavoratori schiavi». Come un attuale presidente di Regione, non molto tempo fa, ha detto: «L'arbitrato è una pistola puntata alla testa dei lavoratori».

le ragioni che hanno condotto alla frequente presenza di deviazioni di carattere violento, non ci si possa poi stupire se qualcuno auspica che

Aule parlamentari, che si è già consistentemente svolto; tuttavia, nel momento in cui c'è l'occasione di svolgere un dibattito in sede parlamentare noto molte assenze, magari proprio di molti di coloro che rivendicavano un dibattito doveroso

Normalmente consentono. In ogni modo, non è mia intenzione aggiungere polemica a polemica. Vorrei soltanto

Di quel tempo egli ricorda in particolare quanto fosse necessario lo Statuto per porre fine alle terribili discriminazioni che, impedendo l'esercizio delle libertà sindacali nei posti di lavoro, tenevano i lavoratori in uno stato di soggezione e di assoluta subordinazione nei confronti degli imprenditori, e usa a simbolo di queste discriminazioni le schedature, così ricorrenti in quel tempo. Ce ne sono alcune, che egli rammenta, particolarmente significative: c'è un terribile lavoratore definito «di tendenza leniniana», che nel 1968 ritenne orientato verso il PSU (Partito Socialista Unificato), già PSI; era l'anno in cui io mi iscrivevo a quel partito, e ne ho un ottimo ricordo. proprio per ricordare quel tempo, Giorgio Benvenuto ancora cita Gino Giugni, testimone di un colloquio con Brodolini, poco prima della sua scomparsa, e Brodolini gli raccomanda di seguire attentamente il dibattito in Parlamento con queste parole: «Io non voglio che lo Statuto dei lavoratori diventi lo Statuto dei lavativi». Anche questo è riformismo, cioè la chiave di lettura dello Statuto dei lavoratori. Carlo Donat-Cattin - che continua a seguire, dopo la morte di Brodolini, l'*iter* parlamentare e la prima implementazione dello Statuto, come ricorda Giorgio Benvenuto ricorda Giorgio Benvenuto - aggiunge: «Non hanno capito che in fabbrica ci si va anche per lavorare e bisognerebbe cercare di mettere qualcosa nella legge che orientasse in questo senso». Questi ricordi sono molto indicativi del clima riformista che sostiene lo Statuto dei lavoratori, che non viene compreso altrettanto bene da componenti che non solo non lo votano ma, come dicevo, radicalmente lo contestano (e non riporto citazioni, che ho qui a portata di mano, dalla rivista giuridica vicina alla CGIL). Tutto questo lo ripeto non per riaprire antiche divergenze, ma per sollecitare un modo molto più paziente di ascoltarci reciprocamente e molto più costruttivo di confrontare le nostre reciproche posizioni. Serve aggiustare lo Statuto dei lavoratori? Serve aggiustare quell'impianto? Sempre Giorgio Benvenuto lo afferma in un modo che mi convince molto. Dice: «Nel modo di parlare si è abituati ad affermare: "Bisogna difendere i lavoratori". Si usa e si abusa, per tutte le scelte di politica sindacale, del termine "difendere". Penso che così facendo si finisca per rimanere immobili, si diventi anzi conservatori. Oggi difendere non è più sufficiente: dobbiamo valorizzare il lavoro, la professionalità, il merito, l'impegno». Ho citato Giorgio perché è stato per tanto tempo segretario dell'organizzazione sindacale che più aderì alla UIL. Ha ragione Pietro Ichino quando ricorda che la CISL era solita dire: «Il contratto è il mio Statuto» e che in qualche modo, pur preveggente, quel ragionamento non era tuttavia consono a quel tempo, nel quale esistevano diffusamente quelle discriminazioni che emblematicamente si traducevano anche nelle schedature. Ma proprio il segretario della UIL, nonché, poi, parlamentare della sinistra, dice anche: «Dobbiamo cambiare, e adottare modi con i quali non soltanto affidarci a diritti fondamentali e inderogabili di legge sanzionabili, ma dobbiamo individuare anche una dimensione promozionale dei diritti e ancor più delle tutele che li sostengano e li rendano effettivi nella realtà che cambia». Pensiamo ai diritti fondamentali nel lavoro. Credo che possiamo, insieme, riconoscerli oggi nel diritto alla salute e alla sicurezza nel lavoro, nel diritto alla giusta remunerazione del lavoro, nel diritto alla occupabilità, cioè ad essere posti continuamente nella condizione di essere occupabili. Se noi guardiamo alla norma inderogabile di legge, troviamo alcune opportune disposizioni che vanno probabilmente mantenute, essere modulate quando sono tutele che possono esserlo, che sono già modulate nello Statuto dei lavoratori, ma vediamo come tutto ciò che è sanzionabile è molto insufficiente a rendere effettivi questi diritti, perché pur avendo un impianto normativo così pesante, questi diritti che ho citato non sono così effettivi come tutti insieme credo vorremmo. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nel lavoro, certo, abbiamo definito molti adempimenti che sono sostenuti da adeguate sanzioni, ma avvertiamo il bisogno di aggiungere molta attività promozionale in termini di formazione, informazione e prevenzione. Per quanto riguarda la giusta remunerazione, non ci accontentiamo di ciò che è sanzionabile, cioè del salario definito dal contratto collettivo al quale la giurisprudenza riconosce un'efficacia *erga omnes*,

incorpora anche un elemento fortemente partecipativo del lavoratore al rischio di impresa, non solo per i profili negativi, ma anche per quelli positivi. Se guardiamo al diritto all'occupabilità, pensiamo all'articolo 18, sappiamo quanto esso non difenda per nulla un posto di lavoro quando questo si consuma, e come solo l'investimento nelle conoscenze, l'accesso alla conoscenza, alla competenza, e la possibilità continua ed effettiva di migliorare le proprie conoscenze e competenze definiscano una continuità nel rapporto di lavoro e possa addirittura rovesciare il rapporto di forza fra lavoratore e datore di lavoro, quando il datore di lavoro è indotto non solo a dare un contratto a tempo indeterminato, ma a cercare di fidelizzare quel lavoratore così professionalizzato che appare nel mercato del lavoro più libero dello stesso datore di lavoro nel cercare un'altra un'altra soluzione a lui più consona. Sono casi rari, ovviamente in questo contesto, ma insisto su quanto si riveli necessario lo strumento dell'investimento nelle conoscenze e nelle competenze. lo Statuto dei lavori è un modo per far vivere lo Statuto dei diritti dei lavoratori: non è un modo per

A questi lavori abbiamo già dedicato alcune disposizioni proprio con la legge Biagi: penso alle tutele della maternità o alla norma relativa alla giusta remunerazione del collaboratore a progetto, spesso ancora troppo ineffettiva. Basti vedere le differenze di remunerazione per uno stesso collaboratore, magari anche correttamente tale perché opera in *outbound* in un *call center*, ma che per la stessa prestazione viene retribuito in modo così diverso e talora talora così misero, a mio avviso contravvenendosi a quella che è già una norma di legge. Quelle stesse protezioni possono essere ulteriormente codificate ed estese, così come

grazie allo Statuto dei lavoratori, le parti sociali possono incontrarsi virtuosamente, adattarsi reciprocamente e, molto più effettivamente ed efficacemente, rendere attuali e praticate quelle tutele che rendono effettivi i diritti fondamentali a cui mi riferivo. Questa sussidiarietà verso gli attori sociali è essenzialmente il contenuto del passaggio che questo Governo vorrà proporre: il passaggio a quel maggior riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva nella sua più forte articolazione e nei tanti dualismi che caratterizzano il nostro mercato del lavoro e che si sono fortemente sviluppati dal tempo nel quale l'assetto della produzione, l'organizzazione del mercato del lavoro e le persone in esso attive avevano caratteristiche molto più standardizzate. Oggi, invece, i dualismi sono numerosi, a partire da quello territoriale, che purtroppo si è confermato. E come non pensare a un diritto del lavoro, a una regolazione del lavoro, a un sistema di relazioni industriali che aiutino soprattutto la crescita, in un tempo nel quale questa sarà resa difficile dalle condizioni di Paesi (quelli europei, dell'Europa mediterranea in modo particolare), ove si combinano alto debito pubblico e declino demografico? Tali caratteristiche, invece, si trovano in modo opposto nei Paesi oggi più vitali, che chiamiamo emergenti ma che, in realtà, sono già emersi e che nella ripresa stanno crescendo con un ritmo straordinariamente superiore alla vecchia Europa. Ma come realizzare crescita, e crescita con occupazione? E come organizzare distribuzione equa della ricchezza, una volta che questa si produce attraverso posti di lavoro e salari come dicevo - quanto più ai risultati e agli utili stessi dell'impresa? Queste sono le sfide che abbiamo di fronte, rispetto alle quali le ricette sono tutt'altro che semplici, ma per le quali occorre disponibilità al confronto reciproco, all'ascolto reciproco e disponibilità di tutte le parti sociali a mettersi in a mettersi in discussione e a trovare punti d'incontro. Quando si realizzano accordi, come quello, che io ho apprezzato, di Banca Intesa con le organizzazioni sindacali per assumere 1.000 giovani a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sulla base di un salario di ingresso per un determinato periodo di tempo; quando si realizzasse, come io spero, un accordo a Pomigliano d'Arco per attrarre la produzione della Panda, che il gruppo FIAT ha proposto di localizzare in quella sede, anche rispetto ad altri stabilimenti all'esterno del nostro Paese; quando le parti dovessero realizzare un punto d'incontro e un'adattabilità reciproca, circa tempi e metodi di lavoro e circa l'orario di lavoro, fra le esigenze di competitività, da una parte, e le esigenze di qualità del lavoro e di qualità della vita che il sindacato rappresenta, dall'altra; dovessimo via via veder sviluppare questa capacità in sussidiarietà delle parti di organizzare enti bilaterali per dare valore al lavoro, come strumenti continui, flessibili e adattabili per dare valore al lavoro; allora, noi assisteremmo a a idee in movimento, e non soltanto alla statica strumentazione difensiva, a quella difesa che Giorgio Benvenuto invita a superare con così intensa attività delle istituzioni e delle parti sociali. Io ho proposto che nel Mezzogiorno, in agricoltura ma anche nel turismo, cioè in ambiti produttivi caratterizzati da forte disseminazione dei lavori, si adottino le buone pratiche che in edilizia le parti sociali hanno saputo produrre, diffondendo la bilateralità e organizzandola sistematicamente su base provinciale per sostituire i caporali con intermediari legittimi, trasparenti, rappresentativi, come possono essere i soggetti della rappresentatività. Questo è lo spirito con cui affrontare il percorso di fronte a noi. Nei prossimi giorni il Governo presenterà un piano triennale per il lavoro, cui seguirà il disegno di legge delega circa lo circa lo Statuto dei lavori. Il Governo presenterà questi atti sulla base di una fase di dialogo sociale e di trasparente dibattito parlamentare, perché poi, alla fine, toccherà anche al Parlamento, ovviamente, esprimere le proprie opinioni e il proprio voto su quelle e su altre proposte che sono state presentate, io mi auguro nella direzione di un bene comune che non può non essere ritenuto largamente condiviso.